urgenti e concrete per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale e proroga alcune missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

senatrice Stefani, provi a parlare.

come di un'ipotesi particolarmente drammatica ed insidiosa, al punto da vedere tutti noi minacciati da alcune componenti, che nascono purtroppo

che, come si diceva prima, è particolarmente insidioso. Abbiamo bisogno di uomini e di mezzi, perché il controllo del territorio non può prescindere da un'organizzazione di uomini e di mezzi.

È un problema che deve essere affrontato in maniera sistematica. Per l'ennesima volta, invece, vediamo molte delle tematiche in questione, passate anche al vaglio della Commissione giustizia, di cui faccio parte, affrontate in modo

Come possiamo pensare che il sistema delle Forze dell'ordine possa riuscire a verificare l'attività di ogni singola persona?

in mezzo a tutto questo c'è il problema del terrorismo. E il terrorismo non è il furto di un orologio in un appartamento, non è il furto di un'auto, ma un rischio totale per la nostra collettività.

interna. *Primum vivere, deinde philosophari*, qualcuno aveva anche detto: prima troviamo una sicurezza per i nostri territori, poi possiamo fare anche altri ragionamenti.

e assecondano numerose esigenze di natura sia repressiva sia preventiva, anche se non mancano certo le criticità. Nelle situazioni di emergenza, come quella che l'Italia e l'Europa stanno vivendo, non è mai facile trovare un punto di equilibrio fra le esigenze di sicurezza e la tutela non solo della *privacy*, ma anche delle libertà fondamentali dello Stato di diritto. In tempi ormai lontani, ma di cui molti di noi hanno ancora un drammatico ricordo - mi riferisco agli «anni di piombo» lo Stato riuscì a vincere la sua battaglia senza ricorrere a sistematiche normative emergenziali. Oggi la minaccia è ancora più insidiosa perché abbiamo di fronte un'organizzazione terroristica che si è fatta Stato e che, a causa dei gravissimi errori dell'Occidente, sta espandendo la sua zona di influenza non solo alla Libia, ma a tutto il Maghreb, ossia a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, lucrando sul traffico dei clandestini e facendo proseliti anche nel nostro Paese col fenomeno dei *foreign fighters*. Ma veniamo ad esaminare in dettaglio il decreto-legge che introduce nuove figure di reato, tra le quali l'auto addestramento del terrorista e i viaggi con finalità terroristiche, e aggrava quelle esistenti se commesse in rete. In effetti, oggi il *web* è la modalità più diffusa per il reclutamento e l'ISIS sta dimostrando di essere un abile gestore dei *social network*; quindi è lì che è giusto appuntare maggiormente l'attenzione. C'è però il rischio reale di incorrere in gravi profili di incostituzionalità. Nel disegnare il diritto penale di Internet, infatti, il Governo ha trascurato i principi della tassatività e della materialità della condotta di reato. Il decreto-legge non tipizza, infatti, in maniera sufficientemente puntuale il comportamento vietato al futuro reo, né accerta la pericolosità concreta della condotta, mentre la Costituzione vieta di punire l'intenzione criminosa priva di una sua concreta materialità. Il decreto-legge propone poi le *black list* per i siti in odore di terrorismo per rimuoverne i contenuti illeciti. In questo ambito le misure si presentano deboli perché non distruggono il contenuto illecito ovunque disseminato sul *web*, ma solo quello del sito, né colpiscono in modo sufficientemente forte i terroristi solitari. Il garante Soro, poi, è già intervenuto per dire che questo decreto-legge deroga vistosamente al codice della *privacy* in modo da favorire la raccolta dei dati da parte delle Forze dell'ordine per accertare i reati, obbligando gli operatori di Internet a conservare i dati delle conversazioni e delle navigazioni per allo scopo di indagare su uno spettro amplissimo di reati nei confronti di chiunque e indipendentemente dal sospetto di un reato. Su una parte di questa problematica si è opportunamente fatto un momento di riflessione. Comunque, l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati relativi al traffico telematico e alle chiamate senza risposta non potrà che agevolare la ricostruzione della rete di conoscenze e dei contatti dei sospettati di terrorismo, ed è quindi difficile rinunciarvi. L'altro punto su cui sarebbe necessario riflettere è quello riguardante l'attribuzione alla Procura antimafia anche del ruolo di Procura antiterrorismo. Mafia e terrorismo sono due fenomeni di grandissima rilevanza criminale, ma che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro e che richiedono, quindi, specializzazioni diverse. Metterli insieme, magari aggiungendovi anche competenze specifiche sulla corruzione, significa scadere nella demagogia. Ed è bene ricordare che lo stesso procuratore antimafia Roberti ha detto che occorrerebbe apportare delle sostanziali modifiche al decreto-legge, soprattutto dove non è previsto nelle competenze dei vertici della DNA il potere di coordinamento sui servizi centralizzati di polizia. Lo stesso CSM non ha nascosto le sue perplessità, affermando che nel decreto del Governo non funzionano né i poteri di coordinamento attribuiti all'ufficio di Roberti, né tantomeno la regolamentazione dei rapporti tra la Superprocura e i servizi segreti. Questioni delicate, che determineranno il futuro effettivo di una struttura che da anni i magistrati impegnati nelle indagini sul terrorismo sollecitano, ma che a questo punto potrebbe nascere zoppa. Sarebbe un'occasione mancata che il nostro Paese non si può permettere, soprattutto a fronte del grave allarme internazionale costituito dal terrorismo islamico. Le criticità messe in rilievo sono essenzialmente tre: la prima, come ho già ricordato, riguarda l'effettivo coordinamento che la futura Superprocura antiterrorismo potrà avere nel rapporto con le polizie centrali. Di fatto essa non se ne potrà avvalere direttamente. Ma non basta. Ad aggravare la situazione c'è il capitolo dei futuri rapporti tra la Superprocura e i servizi. Qui, di fatto, l'ufficio di Roberti è tagliato fuori da un'interlocuzione diretta ed effettiva, perché il decreto-legge ha affidato al procuratore generale di Roma il potere di autorizzare sia i futuri colloqui investigativi in carcere, sia il via libera alle intercettazioni preventive. Due "poteri" che il procuratore Roberti rivendica per sé, per evitare che la Superprocura resti un ufficio più di rappresentanza che operativo. Effettivamente, con l'introduzione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo abbiamo davanti un apparente paradosso: esiste la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ma non esistono le Direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo. Un problema funzionale che non può restare irrisolto. Una misura sicuramente giusta è invece il rafforzamento dell'*intelligence* favorendo le operazioni sotto copertura e allargando le garanzie funzionali per gli infiltrati. La legge n. 124 del 2007 proibisce ai nostri 007 di avere rapporti con giornalisti e membri del clero. Un divieto irragionevole che impedisce agli apparati di sicurezza di reclutare come fonte informativa un giornalista di Al Jazeera o l'*imam* di una moschea ufficiale. Ora, almeno, c'è un piccolo passo avanti: quello che consente agli agenti dei servizi di fare colloqui investigativi in carcere, previa autorizzazione. Il decreto-legge contiene anche la proroga dell'"operazione strade sicure", una misura che va nella giusta direzione, ma che richiede, come conseguenza immediata, lo sblocco del *turnover* delle forze di polizia, considerata l'attuale carenza di organico, in quanto la minaccia terroristica è destinata a durare nel tempo e sarebbe assai difficile garantire altrimenti la vigilanza degli obiettivi fissi. Secondo i sindacati di polizia, siamo molto lontani dal miglioramento degli effettivi livelli di sicurezza. Viene facile a questo punto chiedere come mai il Governo non destina almeno una parte del presunto tesoretto trovato tra le righe del Documento di economia e finanza al potenziamento delle Forze dell'ordine, che garantiscono in condizioni difficilissime la sicurezza di tutti in condizioni che definire precarie è un eufemismo.

senza una legge quadro. È vero. Avete appena annunciato che la stiamo dibattendo alla Camera. Ma mi sa che sarà un annuncio secondo la classica "annuncite" renziana su tutto il resto. Quindi, finché non vedremo i fatti, è inutile che ne parliate. Di fatto è da anni che proroghiamo missioni senza una visione strategica - questo sinceramente è alquanto bislacco, visto che parliamo di guerra - e senza coinvolgere il Parlamento. Le spese militari sono le uniche che sono cresciute in questi anni; anni di profonda crisi; e non hanno risolto nulla, mi sembra, ma hanno complicato il quadro internazionale. Mentre spendete cifre esorbitanti e senza criterio, intanto citate i tesoretti. E fate schifo anche in questo, perché siamo in campagna elettorale e ve la volete vendere con i cittadini, come con gli 80 euro. Bene, anche questo è un comportamento indegno, indegno per voi, perché stiamo parlando invece di una questione che parrebbe molto importante, quella del terrorismo, appunto. parliamo di terrorismo. Cosa fa il terrorismo? Lo si sa ed è abbastanza banale come cosa. Nel titolo, dite che questo decreto-legge riguarda misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale. Questo "anche" è molto interessante e vi spiego perché. Il terrorismo diffonde terrore, panico, instabilità; il terrorismo destabilizza e quindi colpisce a sorpresa, senza avviso e senza nessuna previsione, obiettivi sensibili, luoghi pubblici, infrastrutture. Semina il panico e la paura nella vita quotidiana dei cittadini, che si sentono esposti a pericoli mortali. In questi giorni abbiamo sentito del tetto di una scuola che è caduto sugli studenti. In Piemonte, in Provincia di Torino, è morto uno studente, al liceo «Darwin», proprio per un crollo. Sono crollati ponti e strade, nuovi di pacca, appena fatti, appena consegnati. i tribunali, hanno ucciso un giudice in un tribunale, così, senza nessun preavviso, vagando tra l'altro senza nessun controllo all'interno del tribunale. Oggi, tra l'altro ci sono stati cinque feriti al tribunale di Napoli, per i tafferugli dovuti ad una gestione della sicurezza evidentemente inappropriata, fatta così, di corsa, per mettere un tampone.

Non c'è stata nessuna capacità di gestione, perché, se adesso vogliamo, con il ministro Alfano, gestire la sicurezza nei tribunali o in altri luoghi strategici come voi state facendo, mi sembra che fermerete di più la giustizia invece che garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi a me sembra sinceramente che, più che da un terrorismo internazionale, il nostro Paese si debba guardare dal terrore che provocano questo Governo, i Governi precedenti, questa maggioranza e i decreti-legge che votiamo con la fiducia, come probabilmente succederà anche oggi, i quali sono molto più gravi e molto più pericolosi del terrorismo internazionale. Il ministro Alfano, mentre cercava di infilare proprio in questo decreto-legge incostituzionali invasioni della *privacy* dei cittadini tramite virus o *trojan* informatici, si scagliava il giorno prima contro le intercettazioni Ma guarda caso!

non ci sono più servizi. Nella mia città, io vivo in un quartiere dove dobbiamo convivere con un 30-40 per cento di immigrazione e lo dobbiamo fare da soli, abbandonati, con un livello di microcriminalità altissima; i primi a protestare sono proprio gli immigrati regolari che stanno lavorando.

Questo Paese si deve guardare da voi. Volete salvarci? Andatevene. Signora Presidente, siamo in presenza di un provvedimento che chiama in causa un Paese ed una comunità, in un momento di emergenza di emergenza e di grande criticità, in cui la sicurezza di tutti noi è messa a repentaglio da una presenza terroristica che si muove con modalità inusuali. inusuali. La coscienza collettiva e quella di ognuno di noi è chiamata a far fronte ad un fenomeno di terrorismo internazionale che non si muove solo solo in modo assolutamente marginale e con modalità consuete, ma sta mettendo in campo modalità nuove; modalità nuove; mi riferisco soprattutto ad un grande utilizzo dei mezzi di comunicazione, da Internet alla televisione, alle immagini, ai *video* girati che tutti noi abbiamo potuto vedere;

immigrate da Paesi e comunità di cultura islamica, che oggi sentono il richiamo di quelle organizzazioni e di quelle teorie. Contemporaneamente, siamo di fronte al solito dilemma che investe una comunità nel momento in cui decide che è il momento di mettere in campo misure di sicurezza emergenziali, cioè la consapevolezza che in un Paese democratico, in un Paese di diritto avanzato, l'eccessivo ricorso a misure di sicurezza non può non trovare un suo contraltare in una riduzione dei diritti di cittadinanza e dei diritti di libertà. È rispetto a questo equilibrio che siamo costretti, anche in questo caso, a confrontarci. Io ritengo che la misura individuata da questo provvedimento possa essere accettabile rispetto a questo equilibrio, seppure con alcuni elementi di criticità, di cui dirò, su cui credo che l'attenzione di ognuno di noi debba rimanere molto alta.

Fatte queste precisazioni, è indubbio che oggi noi abbiamo la necessità di dotare le nostre istituzioni di strumenti efficaci. Qualcuno ha voluto paragonare la minaccia del Daesh, quello che viene impropriamente definito Stato islamico, alla terribile minaccia per l'ordine internazionale costituita, nel secolo scorso, dal pericolo nazista. È evidente che siamo di fronte ad un fenomeno del tutto diverso da quello, ma è altrettanto evidente che possiamo trovare segni inequivocabili di relazione con quel questo gruppo terroristico, che si autodefinisce Stato, tratta il rapporto tra il potere politico e libertà

alleati - penso ad esempio a Boko Haram - che oggi si trovano in uno stato di privazione del loro diritto all'infanzia, ma che spesso è privazione della libertà e spesso è privazione dell'integrità fisica

penso a quello che sta accadendo ad esempio alle persone omosessuali, sterminate senza pietà nelle zone controllate dal *Daesh*; penso alla minaccia inumana, alle argomentazioni fredde, ciniche e spietate, che i dirigenti e i militanti di questa organizzazione mettono in campo per accompagnare le loro azioni. Noi siamo vicinissimi a questo pericolo. Il fatto che Roma sia stata evocata più di una volta come possibile obiettivo di un'azione terroristica non va considerato solo come una provocazione: siamo in un contesto in cui un pericolo reale è possibile.

che riesce a intervenire su tutto il Pianeta, ma anche con azioni terroristiche messe in campo da gruppi ristrettissimi di persone, spesso da singoli individui o da gruppi composti da poche unità

tipo, le misure di cui stiamo oggi parlando siano poco efficaci. Può darsi che sia così, anzi sicuramente questa frammentazione del pericolo terrorista è un ostacolo alla pianificazione di azioni di prevenzione, di repressione e di contrasto. Da una parte è inevitabile che comunque mettiamo in campo tutte le misure a nostra disposizione; dall'altra parte, è indubbio che alcune delle previsioni contenute in questo decreto-legge tengano conto di questa specificità. Mi riferisco, ad esempio, all'introduzione di quelle nuove fattispecie penali che parlano di addestramento o di arruolamento tramite Internet di queste persone, o addirittura puniscono l'autoaddestramento tramite Internet cioè quella singolarità e quella specificità di persone che, magari dalla periferia di Parigi, di Londra o di un altro Paese europeo, costruiscono una loro presenza

del Governo, nostra e di chi dovrà monitorare l'implementazione di queste previsioni, dovrà essere alta. Mi riferisco al passaggio in cui si introduce come pena accessoria la perdita della potestà genitoriale quando in questa attività è coinvolto un minore.

ora direttamente ad alcuni punti di criticità su cui bisognerà intervenire. L'inserimento del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra i reati ostativi alle misure alternative e ai benefici penitenziari non deve farci dimenticare che la platea di chi è sottoposto all'esclusione da tali benefici deve essere sempre fortemente controllata, monitorata e non eccessivamente perché anche in questo caso stiamo parlando di una sospensione di diritti di garanzia previsti dal nostro ordinamento. Chiudo ricordando il tema, su cui peraltro il Garante della *privacy* ha costruito una serie di argomentazioni non sempre recepite da questo

*(PD)*. Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare i relatori, senatori Vattuone, Ginetti e Maran, per il lavoro svolto nelle Commissioni riunite sul decreto-legge oggi al nostro esame. provvedimento importante perché prevede, in un momento di emergenza nazionale e internazionale, misure urgenti e concrete per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale e proroga alcune missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, selezionando le priorità e

per l'autodeterminazione del popolo Saharawi e sul mantenimento nella zona del cessate il fuoco. Proprio su questo ho presentato un ordine del giorno, assieme a tanti colleghi dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo a dare continuità, già nei prossimi mesi, con ogni possibile sollecitudine, alla partecipazione italiana alla missione Minurso e alle iniziative di sostegno al popolo Saharawi. In quest'Aula della questione Saharawi ne abbiamo già discusso ampiamente nell'aprile 2014 quando fu approvata la mozione 1-00129 (testo 3), a larghissima maggioranza, che chiedeva impegni precisi al Governo in sede europea ed internazionale. È utile tuttavia ricordare che nel 1991, dopo il cessate il fuoco, con la mediazione delle Nazioni Unite, si è pervenuti all'avvio di un processo di pace sostenuto attraverso numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo ancora non raggiunto di far svolgere un *referendum* per l'autodeterminazione del popolo Saharawi. Esattamente per sorvegliare sul cessate il fuoco e presidiare questo processo di pace, il 29 aprile del 1991 fu istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione n. 690, la Minurso, che da subito poté contare su 100 osservatori internazionali. Per citare dati più recenti, nel 2014 era composta da 503 persone provenienti da 33 Paesi, di cui 226 militari e 262 Il nostro Paese è tra i pochissimi ad aver dato continuità alla propria presenza tra i caschi blu fin dagli esordi della missione, assicurando per il periodo 1999-2001 la presidenza della Commissione identificazione, mentre dal settembre 2005 al febbraio 2007 un italiano è stato rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per il Sahara Occidentale e capo della Minurso. Non solo: l'Italia si è da sempre contraddistinta per la significativa presenza di associazioni che un po' in tutte le Regioni hanno instaurato rapporti di amicizia e gemellaggio col popolo Saharawi in esilio a Tindouf nel deserto algerino; grazie all'attività diplomatica svolta dal Fronte Polisario esso è stato destinatario di molti progetti di cooperazione allo sviluppo, di molte iniziative di solidarietà e sostegno concreto e politico da parte di associazioni e comitati della società civile, di migliaia di enti locali, Province e Regioni. progetti finanziati in parte da risorse pubbliche, nella maggior parte da risorse private, tuttavia sempre in modo chiaro, trasparente e documentato, accessibile a tutti coloro che vogliano verificarne la corrispondenza tra obiettivi e risultati. Grazie al ruolo svolto da tavoli istituzionali in raccordo con i coordinamenti sulla cooperazione internazionale, da iniziative parlamentari come l'Intergruppo di amicizia con il popolo Saharawi, al quale da molte legislature aderiscono centinaia fra deputati e senatori di ogni forza politica, è stato possibile stimolare il Parlamento italiano ad assumere ogni volta una posizione coerente con le diverse e numerose risoluzioni delle Nazioni Unite. Avendo la fortuna e l'onore di presiedere in questa legislatura l'Intergruppo parlamentare, voglio dire che, pur comprendendo le ragioni e le motivazioni che i relatori hanno ben chiarito a sostegno di questo provvedimento, interrompere o ridurre l'attività come Paese di sostegno alla Minurso può essere interpretato come una presa di distanza dell'Italia dal processo di pace avviato nel 1991, sempre sostenuto e incoraggiato, allontanandola dall'impegno per una soluzione giusta, equa e negoziata del conflitto nel Sahara Occidentale. Sottolineo inoltre che in quell'area non sono da escludere concreti rischi di ripresa dello scontro tra Regno del tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, a causa del peggioramento della situazione socio-economica, al crescere di una situazione di malessere e di frustrazione che sta aumentando soprattutto tra la componente giovanile dei campi profughi, che può diventare facile preda di falangi dell'ISIS già presenti nel vicino Mali. Sin dalla sua costituzione la Minurso ha avuto un chiaro obiettivo di pace e - voglio sottolinearlo con forza - la sua presenza è fondamentale in un territorio (il Sahara Occidentale) che vede all'ordine del giorno la violazione dei diritti umani. Proprio per questo credo che il Governo dovrebbe agire nelle sedi internazionali per far estendere le sue competenze al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza dei cittadini saharawi. Si tratta d'altronde di una richiesta che proviene da tempo dalla maggioranza degli Stati membri del Consiglio di sicurezza, ad eccezione della Francia, che ha sempre ritenuto che il Marocco, avendo fatto dei passi in avanti su questo tema, sia in grado di vigilare da solo su questo delicato problema, ma la storia ci dice che non è così. Il Marocco ovviamente si è sempre opposto, poiché ritiene che il territorio del Sahara Occidentale ricada sotto la sua sovranità; tale sovranità tuttavia non è mai stata riconosciuta da nessun organo dell'ONU o internazionale, né da alcuno Stato. La repressione, gli arresti arbitrari, le torture ed i processi sommari nel Sahara Occidentale e in Marocco sono documentati da innumerevoli rapporti delle organizzazioni internazionali, Amnesty International, Human Rights Watch, la Fondazione Robert Kennedy e da rapporti prodotti nell'ambito delle attività delle Nazioni Unite. Davanti a questa repressione violenta queste organizzazioni e i difensori Saharawi dei diritti umani si sono sempre rivolti con fiducia alla Minurso, scoprendo - ahinoi - che i caschi blu non avevano alcun mandato per proteggere la popolazione, per garantire il rispetto dei diritti umani, principio fondativo delle stesse Nazioni Unite. È per queste ragioni che l'impegno assunto dal Governo in Commissioni riunite qui in Senato e in Aula alla Camera a valutare l'opportunità di ripristinare le risorse necessarie a dare prosecuzione alla missione e a proseguire l'attività diplomatica per l'ottenimento di una giusta ed equa soluzione al problema del Sahara Occidentale dovrà per noi essere opportunamente integrata con l'estensione al monitoraggio sui diritti umani da parte da parte della Minurso e a rendicontare le attività svolte sui sette impegni assunti nell'aprile scorso dal Governo italiano di fronte a quest'Aula. Invito pertanto in questa sede i Presidenti della Commissioni esteri e diritti umani, assieme ai membri dell'Intergruppo, che rimangono a disposizione, a esercitare fino in fondo il loro ruolo

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi discutiamo si inserisce in un contesto straordinario e ben definito di diritto internazionale. Il fondamento normativo del provvedimento risiede infatti nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata nel settembre dello scorso anno, che tratta delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale causate da atti di terrorismo. Il decreto-legge si colloca quindi all'interno di un ambito ben preciso, che è quello della piena partecipazione dell'Italia all'impegno della comunità internazionale contro la grave minaccia terroristica e risponde ad una richiesta assai netta e dettagliata fatta dalle Nazioni Unite. Le norme sono dunque rette da una filosofia legislativa unitaria, rappresentata dalla tutela della sicurezza dei nostri cittadini attraverso misure di carattere nazionale e internazionale. Quest'obiettivo è ben evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, nella parte in cui afferma che «la lotta al terrorismo va realizzata in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*». Il contesto che si deve affrontare rende cioè essenziale sviluppare una capacità di risposta globale attraverso misure che si muovono sul versante sia interno, sia internazionale. D'altra parte, misure efficaci di contrasto al terrorismo, unitamente alla conferma delle missioni internazionali, cui contribuiscono militari e civili, costituiscono il presupposto affinché il nostro Paese possa assumere la tanto auspicata maggiore centralità nelle relazioni internazionali, in considerazione della nostra proiezione di Paese cerniera tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente e del prestigio guadagnato in tanti teatri di crisi. Dopo tale premessa, entro nel vivo del decreto-legge, che si fonda sostanzialmente su due pilastri: il primo è legato alla repressione diretta, aumentando le pene per i reati con finalità di terrorismo, ed alla prevenzione degli eventuali che possono essere commessi; il secondo è legato al rinnovo delle missioni internazionali. Credo sia giusto e doveroso mandare un messaggio di gratitudine e vicinanza

In relazione alle missioni internazionali, vorrei evidenziare come, nel corso degli anni, la partecipazione delle Forze armate italiane abbia assunto una considerevole importanza. Ai tradizionali impegni di natura prettamente militare, in sinergia con gli interventi di natura civile, le nostre Forze armate e di sicurezza si sono invero fatte carico di una serie di iniziative finalizzate alla ricostruzione del tessuto locale, politico e sociale. Nei mandati delle missioni ONU è sempre più frequente trovare compiti che includono la protezione dei civili, l'assistenza nelle operazioni di disarmo ed il supporto alla realizzazione di un processo democratico. Si è passati, quindi, da semplici operazioni d'ingerenza umanitaria, attraverso l'invio di osservatori internazionali, a missioni di mantenimento della pace (*peace keeping*), di formazione della pace e prevenzione dei conflitti (*peace making*) di costruzione della pace (*peace building*), fino ad arrivare a missioni d'imposizione della pace (*peace enforcement*). Il decreto-legge contiene quindi le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine della partecipazione italiana

e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi); Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa e Repubblica centrafricana). Nel decreto-legge sono previste anche disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. Si tratta della parte che più caratterizza l'impegno italiano nelle missioni internazionali, secondo un modello di cooperazione universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale e noto come «modello Italia». Tale modello allude al fatto che l'intervento di natura civile, finalizzato a portare sollievo, maggiore benessere e prospettive di rispetto dello Stato di diritto alle popolazioni locali, contribuisce anche alla lotta contro il terrorismo, nella misura in cui riesce ad erodere alla base il consenso che lo stesso costruisce sul territorio. È dunque essenziale costruire un rapporto di fiducia e collaborazione con le popolazioni e operare positivamente soprattutto per la ricostruzione di un tessuto economico ed istituzionale sano. Per quanto riguarda l'Iraq, come evidenzia la relazione illustrativa, s'intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente al conflitto scatenato dal terrorismo di matrice islamica e all'esodo di sfollati in alcune regioni del Paese, soprattutto nel Kurdistan iracheno. Si proseguirà l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, imprescindibile fattore identitario di una convivenza multietnica e multireligiosa, sia attraverso competenze italiane d'eccellenza sia con la collaborazione dell'UNESCO. A questo proposito, signora Presidente, ci tengo a sottolineare che non uso i termini che adottiamo nel linguaggio corrente, quali IS, ISIS, ISIL, prendendo atto che si tratta di veri e propri atti di terrorismo, non riferibili ad alcuno Stato riconosciuto. Non ci troviamo, infatti, di fronte ad azioni che fanno capo ad uno Stato, ma di fronte a una modalità terroristica che non può essere identificata né con uno Stato, né con una religione. Il terrorismo di cui parliamo è sovversione sistematica di valori assoluti, di tradizioni religiose, di appartenenze culturali, di diritti e di libertà. Come già trattato ed approfondito nel lavoro delle Commissioni riunite giustizia, esteri e difesa, ribadisco la mia condivisione del provvedimento, anche se l'aver attribuito alla procura antimafia competenze dell'antiterrorismo mi lascia qualche perplessità. Sembra che le stesse perplessità siano condivise anche dal procuratore generale antimafia Roberti, come qualcuno ha ricordato poc'anzi. Condivido le dichiarazioni del collega Giuseppe Esposito, anche nel suo ruolo di vice presidente del Copasir, sulla necessità di rafforzare, non solo con mezzi, ma anche con meritate attenzioni, i nostri servizi di *intelligence*, che così bene hanno saputo lavorare finora. Anticipo la presentazione di un ordine del giorno che avevamo condiviso insieme a numerosi colleghi (ma temo che l'avvicinamento verso il il voto di fiducia vanifichi buona parte dei contenuti): si trattava di una modifica correttiva all'articolo 3. Non posso però sottrarmi dal ringraziare i colleghi Caleo, Cantini, Broglia, Di Biagio, Bilardi, Ceroni, D'Ascola, Battista, Vaccari, Albertini, Gasparri, Divina, Bocca e Bernini, che avevano condiviso con me quest'ordine del giorno. Concludo chiaramente con un ringraziamento e con una valutazione positiva del lavoro svolto dai tre relatori Ginetti, Maran e Vattuone, che hanno saputo illustrare sia in Commissione che in Assemblea i 21 articoli, facendoli emergere nel loro significato ma anche nella loro valenza. Sarà, dunque, sicuramente una condivisione positiva e per questo li ringrazio.

un'Aula forse un po' distratta per il tema, così delicato, che stiamo affrontando all'interno della discussione odierna. Parlare di terrorismo, infatti, vuol dire parlare di qualcosa su cui è necessario essere intransigenti, perché si tratta della sicurezza di tutti noi; vuol dire parlare di tematiche che, all'interno di un mondo globalizzato, rappresentano un problema con cui bisogna confrontarsi, anche perché vi è una minaccia che non è ferma, ma che muta continuamente e che assume forme diverse e una una serie di aspetti e iniziative che possono sembrare, a volte, anche semplici da eseguire, ma che viene difficile magari a tutti noi ipotizzare o solamente pensare.

In questo decreto-legge vi sono alcune disposizioni che migliorano l'impianto normativo complessivo, ma ci sono anche delle carenze e delle lacune che sicuramente devono essere sottolineate. Se riconosciamo che vi sono aspetti positivi - mi riferisco in modo particolare all'articolo 6 e all'articolo 8 è necessario anche dire che si poteva e si doveva fare molto di più. Si poteva fare molto di più per quanto riguarda, ad esempio, mezzi umani e materiali; si poteva fare uno sforzo massiccio, sul modello di altri Paesi europei. Penso alla Francia, che in un solo giorno ha reclutato 2.680 persone e le ha inserite all'interno delle Forze dell'ordine e del mondo dei servizi,

attrezzature moderne, che permettano a chi oggi è in competizione con coloro che ci vogliono distruggere e che vogliono distruggere i valori del mondo occidentale di poter competere alla pari. Purtroppo abbiamo a che fare con dei soggetti che conoscono molto bene l'utilizzo di quelle che una volta venivano definite le nuove tecnologie, ma che sono ormai le tecnologie del quotidiano, della nostra vita comune. Tali

questi stessi mezzi di comunicazione, che oggi sono diffusissimi, forse più dei *media* tradizionali. Oggi per avere una notizia in tempo reale non si guarda più

impedendogli di avere la possibilità di diffondere una serie di messaggi che poi, come dicevo all'inizio, condizionano la nostra vita quotidiana. Il problema di questo decreto-legge è che, come dicevo, pur contenendo norme importanti, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione

se non sempre le tematiche più urgenti sono quelle più importanti. Il Governo passa il suo tempo a rincorrere le tematiche più urgenti, dimenticandosi spesso di affrontare quelle importanti e non sempre poi si ha il tempo per affrontare quelle tematiche importanti che magari non risultano essere in quel momento urgenti, ma che sono contingenti e che non si possono dimenticare. Il *vulnus* di questo decreto-legge è proprio questo e chiudo con un'ultima considerazione. Mi auguro che questo decreto d'urgenza, largamente insufficiente per quanto riguarda

credo sia importante far rilevare a quest'Assemblea e al rappresentante del Governo - e non penso di essere l'unico a farlo - che questo ramo del Parlamento si trova ad esaminare per la seconda volta consecutiva il disegno di legge sulle missioni internazionali dopo averlo ricevuto dalla Camera, e senza la possibilità di dare il proprio contributo, visti i tempi ridotti con cui ci siamo trovati entrambe le volte a discutere il testo. esserci anche questa volta Gruppi dell'opposizione a sostegno dell'impegno internazionale del nostro Paese e che ciò possa dare maggior forza all'approvazione di questo disegno di legge; certo, se venisse posta la questione di fiducia, questo potrebbe venire meno. Voglio fare comunque mie le parole del vice ministro Pistelli, che tempo fa ha ben evidenziato quanto sia importante un ampio consenso parlamentare sulle tematiche internazionali. A conferma di ciò credo che chiunque di noi abbia partecipato a qualche missione all'estero abbia rilevanza di quanto appena detto. Nel presente provvedimento è stata inclusa una parte fondamentale di misure volte a contrastare il terrorismo di matrice internazionale, la cui minaccia è sotto gli occhi di tutti e che abbiamo l'obbligo di contrastare efficacemente. A tal proposito voglio ricordare un'analisi che ho ricevuto oggi da un istituto di sondaggi.

Proprio sulle misure antiterrorismo sono state introdotte alcune modifiche al codice penale, che avrebbero meritato un approfondimento maggiore da parte del Senato, se non altro per consentire eventuali miglioramenti che a mio avviso si potevano apportare. In Commissione abbiamo discusso prevalentemente della parte riguardante l'antiterrorismo. Rilevo che le tematiche riguardanti la giustizia, come avviene spesso durante le discussioni in Aula quando trattiamo questo argomento, pongono riflessioni precise sulle quali è necessario esaminare attentamente le disposizioni di modifica, soprattutto le conseguenze che ne derivano nel nostro ordinamento e la loro applicazione. Confido sia l'ultima volta che questo ramo del Parlamento debba correre senza poter incidere. Voglio però approfittare di questa occasione per evidenziare che solamente apportando alcune modifiche ai Regolamenti parlamentari di Camera e Senato

e oggi è all'opposizione faceva la stessa cosa, e viceversa. Detto ciò, vale la pena sottolineare che sono state introdotte alcune disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, integrazioni delle misure di prevenzione e contrasto alle attività terroristiche. C'è quindi un inasprimento delle pene con un aggravante speciale del reato di istigazione contro la personalità interna e internazionale dello Stato (tra cui quelli con finalità di terrorismo). È presente inoltre un'attenzione

compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, agli Internet*service provider* di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. Al mancato adempimento da parte del *provider* consegue l'interdizione all'accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo. Ecco quindi che non si può non riconoscere che queste misure non possano essere che condivisibili. Così come l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per gli scafisti; misura necessaria per questi criminali, trafficanti umani senza alcuno All'articolo 5, comma 3-*ter*, si autorizza l'Arma dei carabinieri ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi Carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quale volontari nelle Forze armate. Tale disposizione è finalizzata a garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Come evidenziato dal *dossier* del Servizio studi, si ricorda che la disposizione viene dettata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge di stabilità 2015 e comunque nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di *turnover*. Apprezzando quindi quanto è stato fatto, credo si debba dare una risposta a tutte le richieste, che non penso di essere l'unico a ricevere, provenienti da idonei ai concorsi di Polizia di Stato e Guardia di finanza. Spero ci sia anche questa volontà politica per apportare le opportune modifiche legislative al fine di poter fare ulteriori assunzioni nel comparto sicurezza senza indire nuovi concorsi.

che impongono di sottoporre i caricatori all'obbligo di denuncia di detenzione. Ciò equivale a paragonarli o equipararli alle «parti d'arma», novero dal quale sono state escluse con il decreto legislativo n. del 26 ottobre 2010 adottato per recepire la direttiva n. 91/477/CEE. Allo stesso modo, le armi di categoria B7 sono prodotte anche da altri Paesi dell'Unione europea, così come i caricatori, e imporre loro delle limitazioni potrebbe essere visto come un ostacolo alla libera circolazione delle merci e al mercato e causare l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese. La vendita delle armi di tipo B7 rappresenta una voce importante nel comparto armiero italiano, che tra produttori, distributori e dettaglianti impiega decine di migliaia di persone. Non sono un cacciatore (anzi, tutt'altro, sono il contrario) e nemmeno un amante del tiro sportivo, però se questa è veramente una misura necessaria per contrastare il terrorismo, credo sia giusto valutare le possibili conseguenze che tali misure potrebbero arrecare in questo comparto industriale.

posto. Sulla parte riguardante le missioni internazionali, prenderò poco tempo, non tanto perché di minore attenzione, piuttosto perché i contesti dove i nostri militari sono impiegati sono pressoché inalterati, credo che chiunque abbia seguito l'impegno del nostro Paese in questi scenari saprà valutare con senso di responsabilità il presente decreto-legge. Prendo atto che il Governo ha stralciato il comma 2 dell'articolo 13 che era oggetto di un mio ordine del giorno approvato nello scorso decreto-legge missioni: peccato che, nonostante fosse stato approvato, non abbiamo avuto modo di avere in Commissione un resoconto dell'attività di manutenzione delle unità navali cedute dal nostro Governo al Governo libico e dell'addestramento del personale della Guardia costiera libica.

da rilevare che vengono altresì stanziati più di 40 milioni per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale, che deve restare una nostra priorità, e auspico che sotto l'egida delle Nazioni Unite ci possa essere un percorso che porti alla stabilizzazione della Libia. Abbiamo tutti contezza di quanto dobbiamo fare per porre il Mediterraneo al centro delle priorità delle organizzazioni internazionali. l'impegno del personale militare italiano possa riprendere prossimamente all'interno della missione di monitoraggio dell'Unione europea EUMM in Georgia, un Paese che, essendo

mi sono recato in Kosovo, mi sono reso conto che quella missione, sebbene duri dal 1999, ha tutta la sua validità ed è giusto che continui ad esistere. Sono stanziati 1.700.000 euro per la realizzazione di programmi di sminamento umanitario fino al 30 settembre 2015. La stessa cifra è stata stanziata per l'intero 2014...

per i viaggiatori): le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. Signora Presidente, intervengo su questo provvedimento riguardante misure di contrasto e prevenzione delle attività terroristiche (anche se altri temi sono trattati in questo stesso disegno di legge), soprattutto per segnalare una preoccupazione rispetto alla quale vorrei che i rappresentanti del Governo prestassero attenzione. Soprattutto, vorrei che potessimo essere rassicurati circa gli interventi che si stanno programmando. Si parla di prevenzione delle attività terroristiche. Ora, la prevenzione, come sappiamo bene, non riguarda soltanto le misure di modifica delle La prima preoccupazione sulla quale voglio concentrare l'attenzione dell'Aula riguarda le infrastrutture critiche sanitarie.

delittuosi, soprattutto di natura terroristica. La grande attenzione che dovrebbe essere posta in questo momento è alla presenza dentro il piano, che sicuramente il Governo sta mettendo in atto per il contrasto e la prevenzione, di una particolare attenzione nei confronti delle infrastrutture sanitarie. Cosa succede se va in *crash* il sistema tecnologico di un ospedale? Non voglio neanche pensarci, ma sicuramente non soltanto i *monitor* si spengono e si perdono tutte le informazioni che abbiamo a disposizione: da quelli delle sale operatorie a quelli riguardanti la storia clinica dei pazienti. Soprattutto, rischiamo di non potere utilizzare alcune infrastrutture e alcune apparecchiature particolarmente importanti: dalle rianimazioni a quelle salvavita. Rischiamo inoltre di non poter contare su alcuni servizi (ad esempio la raccolta sangue e l'emergenza) che sono importanti,

le infrastrutture sanitarie infrastrutture critiche. Nel 2004, dopo gli eventi del 2001, il Consiglio europeo ha chiesto a tutti gli Stati membri di preparare una strategia per la protezione delle infrastrutture critiche al proprio interno, soprattutto per prevenire possibili attacchi terroristici. Fra le sei tipologie di infrastrutture critiche indicate dal Consiglio europeo ci sono proprio le infrastrutture sanitarie, e sono indicati gli ospedali, i servizi sanitari, i servizi di raccolta sangue, i laboratori analisi, il settore dei prodotti farmaceutici. Fra Fra l'altro, in quella occasione il Consiglio europeo aveva dato una definizione di infrastrutture critiche, ovvero quelle infrastrutture la cui degradazione di fronte ad un evento delittuoso terroristico potrebbe avere un serio impatto sulla sicurezza e sul benessere degli europei e sul funzionamento efficace dei Governi e degli Stati membri. si tratti di un tema sul quale non possiamo non tenere alta l'attenzione. Io immagino che i programmi che si stanno approntando in questo momento a livello nazionale tengano conto della necessità di avere un piano per la salvaguardia delle infrastrutture della sanità: da quelle che garantiscono la fornitura dell'energia e delle telecomunicazioni alle *information technology* e *communication*. consapevoli dei rischi che si stanno correndo in questi ultimi mesi, una ricerca condotta recentemente dà elementi di rassicurazione e di preoccupazione. in pochi minuti, di ricordare che una società di ricerca e consulenza strategica (in particolare nella progettualità ICT), la Netics, proprio a fine 2014 ha svolto un'indagine a campione su 65 aziende sanitarie, per capire qual è la situazione relativa alla loro sicurezza informatica (la sicurezza fisica, logistica e funzionale riguarda solo un aspetto della sicurezza che dovrebbe essere garantita dalla sanità). dalla sanità). Ci sono alcuni elementi positivi, perché si rileva che, nel 76 per cento delle aziende sanitarie ospedaliere intervistate, il responsabile dichiara che la situazione è sotto controllo e si è in grado di affrontare qualunque evento terroristico o comunque qualunque evento delittuoso. Ma il problema è che il 24 per cento delle aziende, che si concentra soprattutto nel Mezzogiorno, sottovaluta il problema oppure dichiara apertamente l'impossibilità ad intervenire per la messa in sicurezza anche solo dei *server*, degli apparati

si verifica. Ma, di fronte a provvedimenti che cercano di prevenire e contrastare i danni connessi ad eventi terroristici, non possiamo trascurare la necessità di prestare particolare attenzione anche a queste infrastrutture. Fra l'altro, purtroppo risulta che le aziende italiane effettuano un vero *assestment* del rischio

perché vorrei che fosse dedicata particolare attenzione a verificare cosa si sta facendo in questo momento per contrastare i rischi che possono derivare da un degrado del sistema nel settore sanitario. E, se necessario, occorre potenziare questa attività, chiedendo a tutte le Regioni di avere un piano specifico per la salvaguardia delle infrastrutture e per la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali.

ci pone dei temi con un approccio disordinato. Si tratta di temi che richiederebbero una riflessione approfondita,

stancamente rinnoviamo le nostre missioni e costosamente ci accolliamo nuovi e più profondi fallimenti.

sulla scena e i riflettori si sono lentamente spostati, perché noi ci muoviamo sempre su messaggi di natura mediatica. Le elezioni svoltesi in Afghanistan non hanno affatto risolto i problemi che riguardano uno Stato all'interno del quale vi sono dei conflitti di natura etnica, dove la volontà di creare un Governo di unità nazionale si è scontrata comunque con la forte presenza di forze conflittuali e nel

come - ad esempio - il diritto ad essere interrogati in carcere solo ed esclusivamente se assistiti.

operazioni, invece di affrontare i problemi nel merito e nel contenuto in modo sistematico, si passa al concetto che il diritto costa troppo e, quindi, si riduce. E questo succede dappertutto:

punto per punto, se non - come diceva il senatore Battista - missione per missione, quanto meno i princìpi fondamentali: questo è l'aspetto

Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, i recenti episodi avvenuti in Europa ed in Tunisia rivelano la necessità e l'urgenza di intervenire per contrastare fenomeni che possono incidere sulla sicurezza del nostro Paese, oltre che sulla stabilità di molti Paesi dell'area mediterranea. Quanto accaduto testimonia non solo l'utilità di mantenere le missioni internazionali, ma la necessità, di fronte alle serie e concrete minacce, di porre un freno ai continui tagli al comparto difesa e sicurezza. Mai come in questo momento storico è necessario avere Forze armate efficienti, professionali e ben equipaggiate. Il nemico è alle porte e non è più tempo di antimilitarismo ideologico, tanto più che parte della politica estera del nostro Paese viene svolta anche attraverso il proficuo impegno delle Forze armate. Ciò detto, il provvedimento in esame, che vuole essere un tentativo di porre un argine normativo alle minacce del terrorismo, risulta essere un miscuglio composito di misure eterogenee. Oltre al consueto rifinanziamento delle missioni, vi è contenuta una serie di norme che riguardano appunto la lotta al terrorismo, anche di matrice internazionale, con interventi sul codice penale e misure specifiche per colpire reclutatori e reclutati, prevedendo nuove pene e nuove sanzioni. istituita la procura nazionale antiterrorismo, accorpata però alla procura nazionale antimafia, non comprendendosi tuttavia la ragionevolezza di tale unificazione, trattandosi di due fenomeni, mafia e terrorismo internazionale, completamente diversi. Si prevede poi l'operazione «Strade sicure», con 4.800 militari che saranno impegnati a supporto delle forze di polizia sul territorio: ottima misura che, però, quando fu introdotta dal centrodestra, dall'altra parte si levò alta l'accusa di voler militarizzare il Paese. Fa piacere oggi constatare che il Governo di sinistra voglia addirittura implementarla. Di rilievo è l'avere previsto una maggiore tutela funzionale per il personale dei servizi di informazione, con la possibilità anche di eseguire colloqui investigativi in carcere finalizzati alla lotta al terrorismo. A tal proposito, crediamo sia utile sottolineare la cruciale opera dei servizi di sicurezza in funzione di prevenzione, dovendosi abbandonare, una volta per tutte, gli stereotipi ed i pregiudizi nei confronti di apparati fondamentali per la sicurezza dello Stato che hanno, però, il difetto di non poter pubblicizzare gli eventuali successi riportati sul campo a difesa della democrazia, della nostra sicurezza e di quella dei nostri contingenti militari impegnati all'estero. In tale contesto, risulta inconcepibile che, a fronte di nuove funzioni attribuite ai servizi di informazione, Forza Italia continui ad essere esclusa, sino ad oggi, dall'organismo parlamentare di controllo. Seguitare a lasciare fuori una forza politica che rappresenta milioni di cittadini appare una risibile forzatura, avendo il nostro Gruppo offerto una soluzione praticabile che forse andrebbe presa in considerazione. In caso contrario, si denoterebbe un'estrema mancanza di sensibilità per un elementare esercizio di opportunità politica, oltre che di stile. il mondo, purtroppo, è in subbuglio, tormentato da tensioni e conflitti con un'Europa che presenta scenari che sembravano relegati ormai nei libri di storia. Nel nostro Paese si rende effettivamente necessaria una opportuna azione di prevenzione da possibili, inquietanti situazioni che giungono dall'area mediterranea, per le quali si ha però l'impressione che non vi sia piena consapevolezza, soprattutto da parte dell'Unione europea. D'altra canto, Unione europea e NATO hanno deciso, sinora, di volgere più l'attenzione verso la frontiera orientale dell'Europa, come peraltro confermato di recente dal Segretario Generale della NATO proprio nel corso di un'audizione in Senato. Diventa, pertanto, urgente da parte del nostro Governo far comprendere con più energia che la vera minaccia arriva dal fronte Sud, dove si gioca la partita cruciale per la sicurezza non solo del nostro Paese, ma dell'intera Europa, la quale non può continuare imperterrita a voltarsi dall'altra parte. È complice certamente il nostro Governo che, nel favoloso e indimenticabile semestre europeo a guida italiana, non ha promosso alcuna iniziativa utile a sollecitare i *partner* europei ad assumere iniziative e e responsabilità su tale rilevantissimo tema. E sul *caos* libico, da cui arrivano le potenziali minacce, registriamo ancora la colpevole inattività di questo Governo, nonostante da molto tempo l'Italia avesse ricevuto mandato ufficioso dagli alleati ad occuparsi della questione libica. Ad averlo imposto erano le ragioni storiche di potenza *ex* coloniale, quelle geografiche ed il fatto che, forse, comprendiamo quel Paese meglio di altri, grazie alla nostra diplomazia e al brillante lavoro dei nostri apparati di informazione. Eppure, l'Esecutivo Renzi non ha mosso un dito allorquando il Governo legittimo è stato costretto a fuggire a Tobruk. Non un dito ha mosso la Francia, che pure è la responsabile principale di quel *caos*. Ancora oggi, però, si balbetta, in attesa che si risolva positivamente l'azione diplomatica dell'Alto rappresentante dell'ONU, Bernardino Leon. Questi, però, deve fare i conti con una miriade di "gufi", tanto cari al nostro caro *Premier*, armati sino ai denti. Lo stesso Leon, nelle scorse settimane, aveva suggerito all'Europa e all'Italia di organizzare, intanto, un blocco navale davanti le coste libiche, per prevenire l'arrivo di armi via mare per quanto ci riguarda, bloccare le partenze e la non più tollerabile invasione delle nostre coste. Ma, da tale misura, che poteva essere efficace, e per noi doverosa, non avendo la caratura economica e sociale per fare fronte da soli alle disgrazie di un intero continente, Governo ed Unione europea hanno preso subito le distanze. Si rimane inerti, piuttosto che dare un segnale di Paese serio e di Europa unita contro le organizzazioni criminali che, attraverso la tratta, finanziano il terrorismo. L'unica azione di prevenzione messa in campo dal nostro Paese, inserita nel decreto-legge in esame con quattro soldi di finanziamento, rimane l'operazione «Mare sicuro», per la quale siamo grati alla ministra Pinotti e al sottosegretario Rossi. Che ben vengano controlli più accurati per prevenire attacchi a naviglio occidentale, oltre che per tutelare i nostri interessi e la nostra sicurezza. Vorremmo, però, capire meglio i contorni di questa operazione, che si è trasformata in corso d'opera da esercitazione a pattugliamento del Mediterraneo centrale. Fino a quando, sottosegretario Rossi? Con la bella stagione e in attesa che si assumano altre iniziative, l'operazione potrebbe trasformarsi in una nuova Mare nostrum, che fu - come sappiamo - un successo sul piano umanitario, ma un fallimento su quello della prevenzione e un costoso e pericoloso volano che ha incentivato le organizzazioni criminali impegnate nella tratta. Per carità, siamo tutti contenti quando si salvano vite umane. Oggi, però, più che mai abbiamo il dovere di coniugare l'accoglienza con le esigenze della nostra sicurezza e nessuno può escludere, tanto meno questo Governo degli *spot*, che tra i migranti non si infiltrino terroristi, anche pochi, un rischio che già molte procure reputano serio e alto. Intanto, con un'Unione europea lenta e sorda nel comprendere la gravità del fenomeno, le misure inserite nel decreto-legge cercano di porre un ostacolo alle nuove minacce. Ma in concreto, probabilmente poca forza deterrente, perché contrastare con il codice penale le intenzioni di chi ha voglia di farsi saltare in aria, di chi ama la morte più di quanto noi amiamo la vita, sembra esercizio arduo. Forse sarebbe stato più conducente investire qualche soldo in più sulla prevenzione, sulla sicurezza interna, pensando a nuove assunzioni o a sbloccare il *turnover*, investendo, insomma, su risorse umane e addestramento delle Forze dell'ordine. Viceversa, gli organici si accingono ad essere ulteriormente svuotati in tante città italiane per l'organizzazione di Expo e del Giubileo, lasciando quindi scoperte importanti aree del Paese, con la minaccia del terrorismo alle porte. Allora, ineffabile Governo, è in ballo la sicurezza degli italiani e i vostri *spot* hanno francamente stancato. Tutte le misure annunciate a difesa di obiettivi sensibili sono frutto di ridicola propaganda e non trovano applicazione, perché mancano gli uomini e i mezzi. Le stazioni e gli aeroporti (compreso Fiumicino) sono privi dei più elementari controlli, e non certo per colpa delle Forze dell'ordine. Mentre si vara questo decreto-legge, il Governo chiude decine di commissariati ed i sindacati di polizia lamentano il mancato aggiornamento professionale per la lotta al terrorismo. Allora, piuttosto che annunciare tesoretti da un miliardo e mezzo da spendere in elargizioni pre-elettorali, come con gli 80 euro in occasione delle elezioni europee, pensi il *Premier* a ridurre il carico fiscale ed utilizzi eventualmente questa presunta somma intervenendo anche sul comparto difesa e sicurezza. Viceversa, facciamo tanti cari auguri non al Presidente del Consiglio, ma ai cittadini italiani che non hanno proprio di che stare sereni con questo Governo! Il rifinanziamento delle missioni, signora Presidente, certamente non è uno spreco di denaro, ma uno strumento prezioso per quei Paesi e quelle popolazioni colpite da conflitti, cui i nostri soldati danno un contributo primario in termini di impegno e sacrificio per la pace. Auspichiamo, tuttavia, che, nel prossimo futuro, tali missioni siano più ponderate, nel senso che, a volte, sembra che il nostro Paese segua solo le scelte altrui: una volta Cameron; una volta, purtroppo, il debole Governo dell'epoca, reso ancor più debole dalle iniziative del Presidente della Repubblica, ascoltò e non seppe resistere alle sollecitazioni di chi oggi, da senatore a vita, gioca allo scaricabarile. Il Governo valuti, una volta e per sempre, se le missioni coincidono con i nostri interessi strategici, evitando di assecondare scelte inadeguate, le cui conseguenze poi ci investono da vicino. Con amarezza, oggi paghiamo il prezzo del pressappochismo e l'inadeguatezza delle Cancellerie di mezzo mondo, costretti costretti a fare i conti con la più grave minaccia agli equilibri internazionali che, attraverso la Libia, continua la sua marcia di avvicinamento al nostro Paese. Concludo, signora Presidente, con due parole sulla vicenda dei due marò. Ufficialmente siamo fermi al ministro degli esteri Mogherini che, un anno fa circa, esordiva nel suo nuovo ruolo, annunciando elegantemente elegantemente alla Commissione difesa del Senato, prima ancora che alla stampa, che si stava per dare corso all'arbitrato internazionale. In più, su proposta del presidente Casini, si acconsentiva a coinvolgere le opposizioni. Naturalmente, non era vero niente: né l'arbitrato, né l'opportuno coinvolgimento delle opposizioni. Da

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, i più recenti fatti accaduti in Europa e in alcuni Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa hanno evidenziato l'espandersi della minaccia terroristica di matrice jihadista. Di fronte al mondo, all'Occidente, all'Europa, c'è una minaccia terribile con la quale confrontarsi unendo le forze e senza cadere nel gioco della paura che, con ogni mezzo ed in particolare con brutalità assoluta, il terrorismo mette in campo per renderci deboli e indifesi. Combattere la loro strategia comunicativa fondata sulla paura e sull'incutere terrore, senza far venir meno o anche solo attenuare il vincolo assoluto di ogni democrazia, cioè sicurezza e libertà, è la priorità assoluta. Varie sono le leve che vanno mosse, avendo però sempre forte ed indissolubile quel binomio (sicurezza-libertà) e i valori, i principi i vincoli della nostra Carta costituzionale. Una di queste prime leve, che lo stesso decreto-legge che stiamo discutendo pone, è certamente una sempre più adeguata politica di prevenzione e di tutela dalle minacce terroristiche: prevenzione che deve essere effettuata non solo sul piano interno, ma anche su quello internazionale, con particolare riferimento ai territori con maggiore criticità, come veniva detto anche questa mattina. Il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi, oltre ad essere la risposta prioritaria per combattere il terrorismo nelle sue varie forme e articolazioni, acquisisce sempre di più anche una funzione di carattere preventivo e diviene un elemento essenziale di politica estera, con positivi riflessi anche sulla sicurezza dei cittadini. Il contrasto al terrorismo necessita, infatti, di un approccio concreto, responsabile e globale alle questioni che esso pone, attraverso misure tese a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione del fenomeno non solo all'interno del nostro Paese, ma anche tramite la partecipazione a missioni internazionali che rispondano alle medesime finalità. E il provvedimento oggi all'esame dell'Aula contiene proprio disposizioni necessarie ed urgenti, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare la crescita di un terrorismo che, specie negli ultimi tempi,

che coinvolge tutte le dinamiche della globalizzazione, mettendo alla prova - come dicevo - le capacità degli Stati democratici di saper garantire sicurezza e libertà, accoglienza e integrazione, laicità delle istituzioni e libertà di culto, traendo forza anche dalla straordinaria capacità delle religioni di creare solidarietà, coesione e sussidiarietà. Allo stato, la minaccia terroristica per il nostro continente, più che da organizzazioni strutturate, proviene da un variegato mondo di fanatici, fatto di lupi solitari e professionisti della guerra rientrati dai fronti della *jihad*.

In questo contesto, diventa dunque indifferibile completare il quadro normativo vigente - obiettivo cui tende il decreto-legge in discussione - introducendo misure adeguate e selettive capaci di prevenire il rafforzamento delle organizzazioni terroristiche e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento di attentati anche nel territorio nazionale. Sono pienamente convinta che l'Italia, che rientra tra i potenziali obiettivi dell'azione terroristica, in virtù sia della sua partecipazione alla coalizione internazionale contro l'IS che della sua centralità per il mondo cristiano, saprà giocare un ruolo fondamentale nelle stesse sfide importantissime che impegnano i musulmani d'Europa e di tutto il mondo, che non si rassegnano al fanatismo apparentemente e infondatamente basato sulla religione. Per questo non solo sono inaccettabili in sé le "teorie" che attribuiscono colpe e responsabilità ai migranti - quelle migliaia di uomini, donne e bambini mossi dalla volontà e dalla necessità di fuggire da guerre e violenze - ma esse indeboliscono anche oggettivamente, tutta strumentale alla sola battaglia del nostro "cortile" di casa, lo schieramento largo e unitario che andrebbe messo in campo per battere davvero il terrorismo e difendere il nostro Paese. Dobbiamo muovere con convinzione verso politiche inclusive che tendano a depotenziare quelle situazioni che possano, in qualche modo, alimentare scelte estremiste. Nella lotta al terrorismo, però, sono altresì importanti una rafforzata cooperazione tra agenzie d'*intelligence* e forze di polizia europee, nonché misure normative che accrescano le capacità d'intervento sul fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*, così come appunto fa il decreto-legge. La domanda che ci poniamo e ci siamo posti è, infatti, come i tradizionali metodi d'indagine e di contrasto al terrorismo possano combattere e contrastare l'odierno terrorismo. I più recenti attentati che hanno coinvolto Paesi occidentali sono stati posti in essere da soggetti non appartenenti strutturalmente ad organizzazioni terroristiche, ma che ad esse si sono ispirati (Al-Qaeda o IS). o IS). Come anche altri hanno detto, ciò rende molto più complicata 1'attività di contrasto e prevenzione e, proprio per questo, diviene fondamentale il contributo che l'*intelligence* è chiamata a dare e a cui il decreto-legge assegna nuovi strumenti. Allo stesso modo, se teniamo conto che abbiamo procure che tra di loro a volte non parlano e che talvolta non riusciamo ad avere neanche le stesse tipologie di trattamento per i medesimi reati, vediamo che, allora, la creazione di un coordinamento d'indagine - l'antiterrorismo che si unisce all'antimafia - può essere veramente per noi molto importante. sono nella prospettiva della coerenza con il più avanzato diritto internazionale le disposizioni contenute nel decreto-legge, volte a dare completa attuazione anche alla risoluzione n. 2178 del settembre 2014 (come ricordava questa mattina il senatore Tonini). Con queste norme - vale la pena ricordarlo - l'ONU obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici anche in territorio estero, consistenti talvolta nell'attività che i *foreign fighters* pongono in essere per affiancare conflitti armati con gruppi e organizzazioni di matrice terroristica. In questo senso è rilevante l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa nel codice penale, quella di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, che punisce con la reclusione da cinque a otto anni anche chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo. Allo stesso modo è importante la punibilità di colui che addestra al compimento di attività terroristiche, quanto di colui che viene addestrato e di colui che acquisisce, anche autonomamente, le le istruzioni per il compimento di atti terroristici, prevedendo un'aggravante nel caso in cui tali delitti siano compiuti avvalendosi di strumenti telematici. ciò è tanto più importante in quanto i fatti recenti ci hanno dato la dimostrazione dell'esistenza di soggetti che davanti al *web*, a casa propria, imparano a mettersi le bombe addosso e pure a farle prima di indossarle, escono escono di casa e, in piena città - come è accaduto a Milano nell'ottobre del 2009 - vanno in una caserma di bersaglieri e provano a farsi saltare in aria. Oggi, quindi, convertendo il decreto-legge in esame, cerchiamo di introdurre in via definitiva una disposizione che punisce anche questo tipo di condotta, prima difficilmente perseguibile. In sintesi, il provvedimento in esame - a mio giudizio e a giudizio del Partito Democratico - fornisce il giusto approccio alla complessità del contrasto al fenomeno terroristico. Ma è anche fondamentale che il decreto-legge non sia unicamente rivolto a rafforzare la normativa penale, sostanziale e processuale in materia di terrorismo internazionale, ma consenta la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione, allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace. Anche se ogni semestre lo affrontiamo, non si tratta di un argomento normale, di una mera ritualità e formalità. Ogni volta abbiamo, infatti, la possibilità di discutere sul contenuto delle missioni, sulla coerenza delle stesse e sul ruolo della cooperazione. L'importante - credo - è riaffermare sempre il principio e il valore delle missioni e della cooperazione. Nel caso specifico delle proroghe, sarebbe stato sufficiente far riferimento alla necessità del Paese di partecipare alla coalizione anti-IS, oppure alla novità della partecipazione di personale militare alla nuova missione della NATO in Afghanistan. Basterebbe nominare solo questi casi per favorire il voto. come Partito Democratico, abbiamo voluto approfondire il ruolo primario dell'Italia all'interno di queste missioni, la nostra partecipazione attiva alla comunità internazionale e, quindi, la credibilità del Paese, la preparazione delle nostre Forze armate, la capacità dell'Italia, ma anche la coerenza delle missioni con le priorità della politica estera italiana e della comunità internazionale. In conclusione, siamo tutti e tutte chiamati a partecipare al mondo che verrà e il nostro Paese, da sempre porta del Mediterraneo, avrà maggiori capacità di garantire la sicurezza dei cittadini quanto più saprà farsi protagonista nei processi di pace e di modernizzazione, sviluppo e democrazia. L'Europa è chiamata a misurare le proprie capacità di influenza politica e culturale per rispondere al terrorismo senza - lo ripeto - limitazioni delle libertà fondamentali, ma investendo sui punti di forza della democrazia. Ed è in questa direzione che passi ulteriori si potranno compiere grazie anche al merito del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea.

una posizione di totale contrarietà alle misure contenute nel decreto-legge. Su questa materia, infatti, non si deve mai smettere di riflettere e di accettare anche punti di vista diversi,

rispondere allestendo gli strumenti più adeguati e manifestando anche la disponibilità a sostenere dei costi.

accettazione degli effetti determinati dalle nuove norme introdotte nel nostro ordinamento. Gli strumenti messi in campo attraverso questo decreto-legge puntano a rendere più efficace l'azione di contrasto e di prevenzione, innanzitutto mediante l'allestimento di uno punto centrale di coordinamento. La procura nazionale antimafia diventa anche procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mettendoci nella condizione di poter interagire con i nostri *partner* europei, di poter scambiare velocemente ed efficacemente ogni utile informazione, di poter coordinare il lavoro delle nostre procure, tanto da intervenire tempestivamente per adottare tutte le misure necessarie ad evitare atti di terrorismo che possano mettere in discussione la sicurezza nel nostro Paese. Quelle norme devono, oggi, sostenere il lavoro gravoso della magistratura e delle forze di polizia, alle quali non mancherà mai il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, anche in condizioni di difficoltà.

come riconosciuto da tutti i nostri alleati e dai nostri *partner* europei ed internazionali. Con il provvedimento in esame intendiamo anche segnalare con forza una questione politica che non può essere elusa; vale a dire la necessità di sviluppare una politica comune europea, più capace di pronunciare un protagonismo in grado di eliminare quei focolai di conflitto che alimentano il terrorismo internazionale e quelle iniziative tese ad impedire la radicalizzazione delle posizioni, che costituisce la premessa o quel brodo di coltura molto utile

essere presente ed attuale, hanno sviluppato ogni utile iniziativa per aggiornare il quadro degli obiettivi sensibili presenti nel territorio nazionale. Da questo punto di vista non solo accogliamo le indicazioni, i suggerimenti e le critiche emerse anche in questo dibattito, ma anche le indicazioni molto utili e pertinenti tese a rafforzare e migliorare il nostro sistema di difesa e di presidio delle funzioni fondamentali dello Stato.

Qualcuno ha messo in discussione il fatto che il Governo voglia portare a compimento l'emanazione e l'approvazione della legge quadro. Ribadisco in questa sede l'impegno continuo e fattivo che il Governo sta portando la Commissione difesa della Camera per giungere quanto prima all'approvazione di una legge quadro che consenta di scindere l'esame delle singole missioni dall'esame di carattere finanziario.

a quanto individuato con questo provvedimento in termini di razionalizzazione delle missioni all'estero, che ha comportato la chiusura di certe missioni e una riduzione della spesa della Difesa di circa il 10 per cento. Il terzo punto, tenuto conto del

3.400 uomini delle Forze armate impiegati sul territorio, con un incremento di 1.800 uomini. Circa 600 uomini aggiuntivi ai 1.800 nell'ambito

di sicurezza nel nostro territorio. Ricordo, proprio perché qualcuno lo ha ribadito sia in senso positivo che in senso negativo, che le nostre Forze armate oggi hanno quella professionalità e potenzialità, già verificata all'estero, per poter intervenire accanto alle forze di polizia in termini di potenziamento e controllo dei punti sensibili. Concludo prendendo spunto dall'ultimo intervento sulla credibilità del Paese e su come questa credibilità sia affidata anche alle missioni all'estero. Credo che effettivamente un

con qualsiasi divisa, con le stellette e senza, che in ogni momento del loro quotidiano si impegnano al fine di garantire la tutela della sicurezza dei cittadini e di questo Stato.

onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1854, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 7, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito. La seduta è sospesa.

Le dichiarazione finali di voto avranno luogo domani mattina, a partire dalle ore 9,30: la chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 11. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori è stato stabilito che, dopo il voto sulla questione di fiducia, l'Assemblea proseguirà l'esame della ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari.

sulla crisi economica e sociale della Sardegna e sulla banda larga. In concomitanza con la riunione di un Gruppo parlamentare, domani, dalle ore 13 alle ore 15, sono sconvocati i lavori delle Commissioni, con l'eccezione delle Commissioni 1a e 5a. Nella seduta di giovedì 16 aprile, alle ore 12,30, il Ministro della giustizia renderà un'informativa sui tragici fatti avvenuti il 9 aprile scorso presso il Palazzo di giustizia di Milano. Seguirà il sindacato ispettivo. La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 21 aprile, alle ore 11, per l'esame del decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali. Restano fermi gli altri argomenti già previsti, con l'intesa che il voto sul Documento di economia finanza avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Pertanto non si svolgerà il previsto *question time*.

sarebbe stato necessario che il Governo evitasse di porre la fiducia. Su argomenti che riguardano emergenze come il terrorismo e le missioni internazionali sarebbe stato necessario ricercare un consenso maggiore da parte del Governo, dato che sono emergenze che riguardano tutti, nessuno escluso. Oltre tutto, una cosa del genere probabilmente avrebbe dato a tutti la possibilità, da una parte, di dare il proprio contributo per fronteggiare un problema di così dall'altra, di dare anche un appoggio ai nostri soldati nelle missioni internazionali. ho una questione che non voglio tenermi nella mia coscienza, ed è un punto che ho già affrontato in passato. colleghi, un Paese a livello internazionale è preso sul serio se è coerente e se fa seguire i fatti alle parole. Nella vicenda dei marò di parole, anche in quest'Aula, ne abbiamo dette tante, ma di fatti - dispiace dirlo - ne abbiamo messi in atto davvero pochi. Ci siamo lamentati, ma poi non siamo riusciti ad evitare che questa vicenda si trascinasse per anni. Tre Governi - quelli di Monti, di Letta, di Renzi .- si sono impegnati invano. Addirittura l'attuale *Premier* aveva posto la questione in cima alle cose da fare, se è vero, com'è vero, che il suo primo atto fu una telefonata di incoraggiamento, e di impegno, in India ai marò. Più di un anno fa avevo proposto qui in Senato, proprio sul decreto-legge missioni, la sospensione della nostra partecipazione alle missioni internazionali contro la pirateria per protesta contro l'atteggiamento del Governo indiano sul caso dei nostri marò, appunto. Come avevo detto allora, è paradossale che i nostri soldati siano processati per azioni compiute nell'ambito di una missione internazionale, e in quest'Aula molti si erano mostrati d'accordo con me. È passato un anno, la situazione non è cambiata granché e ora in questo provvedimento decidiamo di valutare se interrompere o meno la nostra partecipazione a tale missione alla scadenza del prossimo 30 settembre. Mi sembra davvero poco, e il poco in questione è anche poco serio. Una pressione - come dissi nel febbraio scorso, e i fatti mi hanno dato ragione - si esercita non rinviando, ma assumendo subito una decisione forte e, semmai sospendendola in caso di esito positivo. Quindi, in questo provvedimento sarebbe stato il caso, se non proprio di sospendere subito la nostra partecipazione a quella missione, almeno di mettere nero su bianco una sorta di clausola di salvaguardia. Decidere, cioè, già ora un'eventualità semplice semplice, che a livello internazionale tutti avrebbero compreso: l'interruzione al 30 settembre della nostra partecipazione alla missione contro la pirateria senza il ritorno a casa dei nostri marò. Invece, il Governo ha deciso di utilizzare una formula assolutamente generica, dimostrando ancora una volta che le nostre minacce sono scritte sull'acqua. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Ecco perché almeno quell'articolo avrebbe avuto il mio voto contrario. Ma approfitto del caso dei marò per aprire una riflessione più generale. Ci sarà tempo e modo per approfondire il tema, ma voglio qui ripetere che la nostra partecipazione alle missioni ha un senso solo se ci dà la possibilità di avere un ruolo internazionale di un certo peso. Siamo il secondo o il terzo Paese (sia per uomini sia per risorse) come presenza nelle missioni, ma a questo impegno non corrisponde un peso, se non uguale, almeno conseguente nelle decisioni che si prendono negli organismi internazionali. Questa discrepanza magari in passato era accettabile, visto che i focolai di crisi erano lontani. Ma ora, al di là della beffa dei marò, come dobbiamo comportarci se le crisi più gravi le abbiamo dietro casa? Che atteggiamento dobbiamo avere se gli organismi internazionali, a cominciare dalla NATO, sottovalutano la crisi libica e più in generale l'emergere di califfati nel Nord Africa e in Medio Oriente che ci minacciano e possono esportare il conflitto attraverso il terrorismo anche nel nostro Paese, nelle nostre città? Che senso ha mantenere truppe in giro per il mondo, quando l'Italia è sottoposta ad una vera invasione di immigrati clandestini o profughi che fuggono da guerre che si svolgono a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, quasi nell'indifferenza generale, non solo degli organismi internazionali, ma anche di realtà politiche di cui facciamo parte, come 1'Unione europea, che spesso ci lasciano soli? E di questa condizione il nostro Paese sopporta un costo quotidiano, anche nei fatti di cronaca: assicuriamo la sicurezza magari di qualche tribunale afghano, ma lo Stato non ha gli uomini per garantire quella del tribunale di Milano. Ebbene, io non dico che dobbiamo ritirarci, che non dobbiamo più impegnarci. Tutt'altro. Ma la nostra presenza nelle missioni internazionali deve essere coniugata più che mai, e sicuramente più che in passato, con la nostra politica estera, con i nostri interessi nazionali e in relazione al peso che ci può garantire negli organismi internazionali. Non è più il tempo dì essere presenti sempre e comunque in qualsiasi posto. La crisi economica e le guerre che abbiamo dietro l'angolo hanno fatto venire meno la retorica. Spero che di questi problemi il Governo in futuro si faccia carico, di più e meglio di quanto abbia fatto finora.

in ragione anche della ristrettezza dei tempi concessa alla trattazione, che hanno consentito l'approfondimento di alcune interessanti proposte emendative che avrebbero rappresentato un valore aggiunto per l'intero impianto del provvedimento. Tutto questo in considerazione delle posizioni assunte dalle opposizioni su alcune parti del decreto-legge, che hanno indotto il Governo alla determinazione del voto di fiducia. Non posso condividere la scelta di porre la questione di fiducia che, inevitabilmente, fa decadere tutta la discussione parlamentare. Ecco il valore di questa mia volontà di potere esprimere, in qualche maniera, un giudizio su questo decreto-legge. Una presa d'atto che penalizza, ancora una volta, l'operatività di questo ramo del Parlamento. Tutto questo su un provvedimento vario ed eterogeneo dove confluiscono disposizioni anche delicate, come quelle afferenti il contrasto al terrorismo, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato per l'emersione e il contrasto dello stesso. Argomenti nuovi e sensibili che, per quanto legittimi, meriterebbero a mio parere di essere affrontati in un provvedimento adeguato e diverso da quello attuale. Ma posso comprendere la sussistenza di un'urgenza pratica che potrebbe legittimare la natura *omnibus* del provvedimento. Certamente, il decreto-legge in esame assume una configurazione di maggiore rilevanza in ragione dell'attuale congiuntura storico-strategica nella quale l'impegno internazionale del nostro Paese è rinnovato ed amplificato. Il provvedimento, pertanto, risente di questa rinnovata valorizzazione di cui non si può non tenere conto. Le disposizioni, pertanto, definiscono il ruolo che l'Italia e vuole mantenere nello scenario internazionale, sui piano della cooperazione e del supporto alle iniziative di politica estera e di partecipazione alla stabilizzazione degli scenari geopolitici e internazionali, gli equilibri internazionali presentano una situazione complessa e densa dì nuove sfide derivanti dall'emergere di nuovi focolai di conflitto. Senza trascurare la crescente sfida che le nuove realtà legate al terrorismo internazionale pongono a tutto l'Occidente, e all'Europa in primo luogo, dinanzi alle quali bisogna essere in grado di rimodulare gli strumenti dì confronto e di risposta. Lo scenario che abbiamo davanti è in continua evoluzione e questo comporta inevitabilmente una ridefinizione anche del ruolo dei Paesi che sono i capofila nelle missioni internazionali e, conseguentemente, anche dell'Italia. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Anche perché tutti i cambiamenti in atto richiedono posizioni nette. Personalmente sono convinto - e l'ho sempre affermato - della necessità e dell'opportunità di sostenere la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Ciò non solo per le dinamiche e per gli impegni che derivano dalla nostra appartenenza all'Unione europea e agli organismi internazionali, ma anche in considerazione degli ottimi risultati che i nostri contingenti hanno saputo ottenere nei tanti scenari, con iniziative sul fronte della cooperazione e attività di *peacekeeping* che ci hanno visto impegnati in questi anni. Non dimentico il ruolo rilevante svolto dall'Italia in scenari critici, come quello del Libano, senza trascurare le iniziative diplomatiche orientate alla definizione del dialogo con i Paesi islamici moderati e al rafforzamento del modello nazionale di cooperazione allo sviluppo. sono persuaso della necessità di rafforzare le misure di contrasto al terrorismo, proprio in un momento in cui questo fenomeno vede una recrudescenza su diversi fronti. Come dicevo, il provvedimento interviene su molte tematiche che avrebbero potuto essere migliorate attraverso l'azione emendativa del Senato. Pertanto, questa di oggi si configura come un'occasione persa. Non ritengo sia questa la sede per entrare nel merito di eventuali e decadute proposte emendative, ma invito il Governo e l'Assemblea tutta a riflettere su alcuni aspetti non trattati nel provvedimento, che afferiscono ad esempio a quello che sarà il ruolo del corpo militare della Croce Rossa, validamente e storicamente attivo in aree di crisi e che è oggetto di un'opera di vero e proprio smantellamento di cui non possiamo non tenere conto in questa sede, se ci soffermiamo sulla *ratio* di alcune disposizioni del provvedimento; mi riferisco a quelle afferenti al potenziamento e alla proroga dell'impiego del personale militare in ragione di rinnovate esigenze di sicurezza sul fronte nazionale ed internazionale. Non possiamo non intravedere una sorta di contraddizione tra le ambizioni, legittime, del decreto-legge in esame e taluni risvolti pratici e dannosi di altri provvedimenti. Sarebbe necessaria una maggiore armonizzazione quando ci si trova dinanzi alle potenzialità del nostro Paese sul fronte della sicurezza e su quello degli impegni, che non possono e non devono essere disattesi o sminuiti. Un'armonizzazione che è stata invece registrata, ad esempio, sul fronte del coordinamento delle indagini investigative per i reati collegati al terrorismo, che dimostra come sia efficace adeguare ad un sistema operativo già esistente nuovi ambiti di azione che si adattino ad uno scenario in evoluzione. Le premesse sono certamente lodevoli. Ciò che è mancato si rintraccia nel metodo e nell'accostamento di troppe questioni, la cui delicatezza meritava ben altri approfondimenti. Sono certo che la materia in esame, soprattutto per quanto attiene alla lotta al terrorismo e alle novelle normative, troverà spazio in altre occasioni di approfondimento e mi auguro che il Governo offra degli spunti di riflessione a cui anche il Senato possa partecipare in maniera molto attiva.

sono qui a rappresentare la soppressione del potere di sindacato ispettivo riservato ai senatori. Credo di rappresentare anche le esigenze in ordine a molti altri fatti che sono fatti che sono a mia conoscenza. Sono mesi, diversi mesi, che noi non riceviamo alcuna risposta né alle interpellanze, né alle interrogazioni, men che meno alle interpellanze urgenti con la firma di una quarantina di senatori. Non riesco a capire Non riesco a capire quale sia la differenza tra la Camera dei deputati e il Senato, perché da deputato ho trovato sempre puntuale risposta nel giro di venti o trenta giorni alle interrogazioni;

se dall'evanescenza del Governo, che spesso ha tutto l'interesse a non rispondere, dal fatto che contate quanto il due di briscola - con tutto il rispetto che vi è dovuto perché non fate rispettare le prerogative del Senato e dei senatori, e quindi soggiacete a quello cui *ad nutum* il Presidente del Consiglio ed i vari Ministri cioè se rispondere o non rispondere. E quindi mi chiedo: che dobbiamo fare? Qualche gesto eclatante? Ci dobbiamo vestire da *clown*? Dobbiamo fare lo sciopero della fame? Vi dobbiamo fare una pernacchia per dimostrare che non contate assolutamente niente o dobbiamo smettere di interrogare e di interpellare il Governo? non mi dia la solita risposta di carattere eminentemente burocratico «solleciteremo, vedremo, faremo». Concludo per dire a lei ed anche ai funzionari che io, con altri 35 senatori, ho chiesto al Ministro dell'interno di dire una parola chiara sulla tempistica che riguarda le prossime elezioni provinciali in quei Comuni dove si svolgeranno il 20 aprile. 20 aprile. In questi Comuni, soprattutto in quelli commissariati o quelli in via di scioglimento o sciolti perché i sindaci si sono dimessi, in ottemperanza alla legge regionale, per potersi candidare, vi sono intere comunità che vengono escluse, ancorché da un'elezione indiretta, dalla possibilità di eleggere il presidente della Provincia ed i consiglieri provinciali. Se non riusciamo ad ottenere neanche risposte in ordine ed in merito a problemi di carattere generale e così urgenti, perché il 20 aprile si appresta

ha sollecitato giustamente la risposta che è deprecabile non sia stata data. Ci auguriamo che anche questa sollecitazione la possa far scaturire. **Saluto ad una rappresentanza

La Procura nazionale antimafia ha in questi giorni richiamato l'attenzione su alcune aree interne ad Expo date all'associazione di Oscar Farinetti e al suo Eataly ed ha ravvisato - da quanto ci risulta - un procedimento di affidamento di questi spazi senza bando di gara.

che fa parte del patrimonio economico, ma anche culturale di questa città, il grande mercato dell'ortofrutta,

Una Disneyland che pare sia stata concepita e che si realizzerà anche in questo caso grazie a degli accordi

di mediare con le amministrazioni locali affinché il progetto fosse realizzato e mettendo a disposizione le sole strutture (che penso rimarranno praticamente solo delle colonne con delle tettoie). Questo progetto, che è stato spacciato come grande progetto ecologista, grande progetto che avrebbe promosso il chilometro zero, a nostro avviso non farà altro che perpetrare delle vecchie politiche e delle vecchie dinamiche. Vogliamo quindi chiedere e supportare

che quindi non sono passati tramite un bando di gara, come a dire che le brutte pratiche nazionali si riverberano e continuano a perpetrarsi anche a livello locale, grazie, secondo noi, alla compiacenza di amministrazioni che non hanno certo a cuore il bene comune e lo stop al consumo di suolo, ma che hanno invece a cuore ben altri interessi.

con l'accusa di peculato e corruzione. Ancora una volta un voto di scambio: si scambiano crocette sulla scheda elettorale in cambio di concessioni e di posti di lavoro; una consuetudine che ormai sta diventando nota. Ma non è su questo che vorrei concentrarmi, quanto piuttosto sulle conseguenze pagate dai cittadini quando questi soggetti amministrano. Ad esempio, solo per parlare della cittadina di Marino Laziale, esiste il grande pericolo di una megacolata di cemento in una zona in cui c'è un santuario, il Santuario del Divino amore; poi ci sono problemi di distacchi d'acqua, senza nessun rispetto per la dignità umana, e ancora, una gestione dell'immondizia del tutto

dietro tutte queste opere, visto che ha questo modo di agire. Questo è il punto: la gestione clientelare non solo è un danno nel voto di scambio, ma è un danno anche nella gestione della cosa pubblica perché comporta soprusi per i cittadini.

Gli speculatori all'interno delle pubbliche amministrazioni devono sparire perché vivono sulle spalle degli ignari cittadini; quindi tutto quello che è stato approvato da questo sindaco dovrebbe essere revocato. I nostri consiglieri del Movimento 5 Stelle di Marino hanno sollecitato prefetto e Ministro, ma questo scempio indegno, che vede ormai arrestato ogni giorno un sindaco o un amministratore delle vostre schiere politiche, di destra o di sinistra (per modo di dire), deve finire e tutto quello che hanno compiuto questi

faccio presente - ma lo saprete tutti quello che è successo in queste ore - che trafficanti di esseri umani hanno sparato in aria per riprendersi delle imbarcazioni

come una maggioranza e un Presidente del Consiglio chiedano la fiducia su un argomento delicatissimo, di un'importanza direi quasi vitale per il nostro Paese e per l'Europa, ossia sulle misure antiterrorismo e sulle missioni di pace internazionale. Chiedo scusa per l'utilizzo di questa parola forte: è da «criminali» proporlo, ma è atto ancora più criminale accettare la fiducia su tali argomenti. È vergognoso proporre la fiducia su argomenti che riguardano questioni di antiterrorismo e di missioni di pace internazionali. È criminale non aprire e non discutere su argomenti così delicati all'interno di questa Aula. Io non capisco come si possa essere rappresentante del popolo all'interno di quest'Aula e non avere la dignità di far parlare il Parlamento su argomenti delicatissimi e trovare convergenze nell'interesse del Paese e nell'interesse dei nostri concittadini. Allora, io effettivamente mi trovo in grave difficoltà nell'interrogarmi e chiedere a me stesso se all'interno di questo Parlamento molti dei parlamentari sono solo ed esclusivamente delle comparse che non sanno il significato del ruolo che esercitano. Presidente, la prego di concedermi ancora un minuto per fare l'ultima mia riflessione.

per creare le condizioni di una vivibilità migliore del nostro territorio e del nostro Paese o siamo - mi escludo con gran parte di coloro che fanno parte del mio Gruppo - all'interno di questo Parlamento per per esercitare un ruolo, quello di alzare la mano in un determinato momento perché ci è stato suggerito da qualcuno che non conosce le regole della democrazia? Questo è quello su cui mi interrogo. Mi fa paura vedere dei sapientoni, che portano il bagaglio della propria "cultura" nella difficoltà dei movimenti, non capire che dovrebbero difendere i propri figli creando i presupposti di una vera democrazia. Invece la democrazia qual è? Quella di essere ormai schiavi e servi

n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale